Onorevoli colleghi, come sapete, nella tarda serata di ieri l'incubo del terrorismo fondamentalista è tornato a materializzarsi in Europa, con un barbaro, terribile attentato perpetrato a Manchester, nel corso di un concerto a cui partecipavano numerosi adolescenti e ragazzi; un concerto di un'artista, Ariana Grande, che è amatissima proprio dai più giovani, nel Regno Unito come in Italia e in altri Paesi occidentali; dunque, un attentato che puntava consapevolmente a colpire giovani innocenti nel momento della loro spensieratezza. Il bilancio provvisorio è di 22 morti e di circa 60 feriti e, tra le vittime, ci sono anche molti bambini. Come ha avuto modo di dire poche ore fa il presidente Grasso a Palermo, mentre oggi il Paese è impegnato nel ricordo di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, in un giorno di dolore ma soprattutto di speranza e di unione, colpisce veramente come un pugno la notizia dell'eccidio disumano di persone inermi a Manchester. Tuttavia, lo sgomento non può cedere il posto alla rassegnazione e deve, quindi, essere ribadito l'impegno di tutte le istituzioni, a livello nazionale e internazionale, per prevenire efficacemente e contrastare duramente l'aggressione terroristica, nel rispetto dei valori di libertà e di convivenza che rappresentano le fondamenta delle nostre società. «Noi non cederemo al ricatto della paura», ha ribadito questa mattina il nostro presidente Grasso, ricordando peraltro come l'Italia abbia combattuto per decenni il terrorismo e la mafia con gli strumenti del diritto e della democrazia. E - io dico - riusciremo a farlo - ne sono convinta - anche con i nuovi terroristi. Siamo certi che già la prossima riunione del G7, presieduta dall'Italia, rilancerà, rafforzerà e renderà ancora più concreto il comune impegno contro il terrorismo fondamentalista. Nell'esprimere il profondo cordoglio del Senato della Repubblica per il dolore del popolo britannico e la sincera vicinanza alle famiglie delle giovani vittime e ai numerosi feriti, invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento.

in materia di «Riconoscimento della lingua italiana dei segni» e sui relativi emendamenti e, dunque, non è possibile procedere nella discussione. Inoltre, la Commissione giustizia non ha concluso l'esame del disegno di legge n. 2134 e connessi.

Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, approvato dalla Camera dei deputati a conclusione di un *iter* che ha avuto ad oggetto diverse iniziative convergenti sullo stesso obiettivo, è finalizzato a tutelare e valorizzare alcune aree agricole caratteristiche di particolare rilevanza sotto l'aspetto economico, culturale e ambientale, Tali aree agricole sono ritenute di notevole interesse per il loro valore storico, paesaggistico e di salvaguardia del territorio rurale. Appare necessario ricordare come l'agrumicoltura nel corso dei secoli sia stata caratterizzata da una progressiva crescita, tale da modellare e condizionare la società, il territorio e l'ambiente dove veniva praticata, diventando per estesi comprensori parte integrante con il territorio e le tradizioni popolari. Tuttavia, è altresì necessario sottolineare che un settore che rappresentava una fonte di benessere ha subito dagli anni Sessanta una sempre più accentuata perdita di importanza a causa delle mutate condizioni commerciali, sociali e culturali, da ricondurre a diversi fattori, tra cui i crescenti costi di produzione, le ridotte dimensioni delle aziende e la concorrenza estera sempre più forte e aggressiva. Il risultato di tale processo si è concretato in uno stato di crisi aggravatosi negli ultimi decenni, che ha provocato l'abbandono di quelle aree in cui le condizioni di coltivabilità erano più difficili e onerose, con conseguente impatto negativo a livello sia paesaggistico, che di salvaguardia del territorio e con riflessi anche con riferimento all'abbandono di quelle tradizioni che sono state un punto di forza della cultura italiana. Ed è alla tutela di quelle aree che sono rivolte le disposizioni del presente disegno di legge, finalizzate a contrastare le conseguenze dell'abbandono colturale in quelle particolari zone attraverso azioni di promozione e sostegno a favore dei produttori. Appare di significativo rilievo ricordare che il provvedimento in esame è il frutto di un lungo lavoro istruttorio che trae origine dalle precedenti legislature, con particolare richiamo alle iniziative della legislatura scorsa, a dimostrazione di quanto la rilevanza della problematica e l'esigenza di intervento siano avvertite dalle diverse forze in sede politica e parlamentare. Passando all'illustrazione del testo, il disegno di legge si compone di otto articoli. L'articolo 1 delinea le finalità, con richiamo al particolare pregio degli agrumeti e alla stretta connessione del prodotto con le peculiarità del territorio d'origine. L'articolo 2, avente a oggetto la disciplina degli interventi, rinvia a un decreto ministeriale per l'individuazione dei territori dove sono ubicati gli agrumeti caratteristici, la definizione degli interventi ammessi ai contributi e la determinazione della percentuale dei contributi erogabili. L'articolo 3 prevede la concessione di un contributo a copertura parziale delle spese per il recupero e la salvaguardia degli agrumeti, mentre l'articolo 4 ha a oggetto un contributo unico a copertura parziale delle spese per sostenere il ripristino degli agrumeti abbandonati. L'articolo 5 disciplina l'attuazione degli interventi, prescrivendo la conformità degli stessi alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2 e alla legislazione vigente in materia, nonché alla normativa europea. Per l'assegnazione dei contributi citati, l'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione, diversamente dal testo originario, di 3 milioni di euro per l'anno 2017. L'originario articolo 7 sui consorzi di tutela è abrogato, mentre l'attuale testo disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi, che vede il coinvolgimento delle Regioni, le quali dovranno stabilire l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di recupero e di ripristino, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, la selezione dei progetti e la formazione delle graduatorie in base all'istruttoria svolta dal Comune competente. Infine, l'articolo 8 detta le disposizioni sul regime dei controlli e delle sanzioni, affidandone la definizione delle modalità e lo svolgimento alle Regioni e prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie a proprietari e conduttori, nelle ipotesi sia di parziale realizzazione degli interventi indicati, sia di non realizzazione degli stessi. Al disegno di legge è abbinato l'esame della petizione n. 380, che sollecita un impegno per la difesa della produzione di arance, specie nel Meridione. Sollecito quindi una rapida approvazione, per consentire la fruizione degli stanziamenti nell'anno corrente.

Signora Presidente, senatrici e senatori, il disegno di legge n. 1641, che oggi approda in Aula, dopo diversi tentativi nelle legislature precedenti, è un testo che si pone l'obiettivo di sostenere e tutelare un settore, quello dell'agrumicoltura, molto importante per l'economia e il mantenimento del nostro territorio, soprattutto nelle zone particolarmente vocate a questo tipo di arboricoltura. Tutelare e valorizzare le aree agricole del nostro Paese oggi più che mai è diventata un'opportunità per molti dei nostri giovani che, attraverso nuove forme imprenditoriali agricole, contribuiscono al recupero del territorio. L'agricoltura, negli ultimi anni, complice anche la crisi economica, è stata abbandonata dopo essere stata sfruttata intensamente. In quest'ottica, il provvedimento, che mira a promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici nelle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, rappresenta un aiuto e uno stimolo a quanti oggi in Italia hanno deciso di ritornare a reinvestire nella terra, recuperando colture abbandonate in zone marginali. La presente legislatura, del resto, si è caratterizzata anche per avere scommesso sull'agricoltura come settore determinante per la ripresa economica del Paese e dell'occupazione. Il provvedimento in esame non è che l'ultima di una serie importante di leggi approvate dal Parlamento a tutela e sostegno dell'agricoltura, anche e soprattutto quando questa incontra altri settori, come la cultura, il turismo e l'enogastronomia, che in Italia sono un tutt'uno con il paesaggio coltivato dall'uomo nei secoli. La storia degli agrumi è andata di pari passo con quella dell'uomo, rivestendo nel tempo un forte significato sotto l'aspetto culturale, economico, sociale, mitologico e religioso. Le arance e i limoni sono tra i frutti più noti e apprezzati al mondo, sia per la più facile adattabilità alle diverse condizioni climatico-ambientali che per la versatilità dell'impiego nel settore alimentare e in quello non *food*. Al mondo ci sono 5.000 varietà di agrumi, ma possiamo affermare senza alcun timore di smentita che in Italia troviamo la massima espressione della qualità di questa coltura. Il comparto dell'agrumicoltura, nonostante l'elevatissima qualità del prodotto, ha attraversato negli ultimi anni una profonda crisi economico-strutturale che ha portato a un progressivo abbandono delle coltivazioni e, di conseguenza, a uno spopolamento e un impoverimento del nostro paesaggio agricolo. Se da un lato il provvedimento che ci accingiamo a votare oggi in Assemblea mira al recupero e alla tutela degli agrumeti, dall'altro il dispositivo mette in relazione - a mio parere in modo corretto - le coltivazioni con il valore paesaggistico-culturale dei territori dove sono ubicate. Il paesaggio italiano è il risultato di molti anni di storia in cui civiltà e culture diverse si sono succedute e intersecate nella sua struttura costituendone l'identità culturale. Ciò che distingue la complessità dei caratteri storici del paesaggio italiano rispetto ad altri paesaggi europei sono la molteplicità e la stratificazione delle impronte che le molte civiltà che vi sono susseguite hanno lasciato nel territorio, nelle forme di boschi e campagne. Le civiltà hanno dato alle nostre campagne un grandissimo contributo in termini di specie vegetali, tecniche di coltivazione, modi di captazione e uso dell'acqua, costruzioni e manufatti, tanto da far assumere al paesaggio italiano un valore storico unico e del tutto particolare rispetto agli altri Paesi europei e mondiali. Un chiaro esempio di questo sono i terrazzamenti della costiera amalfitana. In determinate Regioni d'Italia, la coltivazione degli agrumi, oltre a rappresentare una fondamentale fonte di reddito per gli agricoltori, ha prodotto dei paesaggi così unici da rappresentare delle icone di bellezza del nostro Paese. Basti pensare ai limoni del Garda, alla costiera amalfitana o alle aree costiere della Calabria e della Sicilia. Queste unicità paesaggistiche colpirono anche Goethe.

Il paesaggio è così unico e importante da apportare un valore aggiunto e una caratterizzazione alle produzioni agrumicole sia in qualità che in riconoscibilità del prodotto nel mondo. l'importanza e la centralità del paesaggio all'interno del provvedimento attraverso il richiamo alla Convenzione europea del paesaggio, all'articolo 1. La Convenzione europea del paesaggio si prefigge si prefigge di promuovere la protezione, la gestione e la pianificazione dei paesaggi europei e di favorire la cooperazione europea. La Convenzione è stata il primo trattato internazionale esclusivamente dedicato al paesaggio europeo nel suo insieme. Oltre a dare una definizione univoca e condivisa di paesaggio, la Convenzione dispone i provvedimenti in tema di riconoscimento e tutela che gli Stati membri si impegnano ad applicare. ad applicare. Prevede la salvaguardia di tutti i paesaggi, indipendentemente da prestabiliti canoni di bellezza o originalità e include espressamente tutti i tipi di paesaggio. L'elevato valore del nostro paesaggio e l'elevata qualità dei prodotti agrumicoli non sono bastati, però, a contrastare il progressivo abbandono delle campagne a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. L'abbandono delle campagne nelle zone particolarmente vocate alla coltivazione degli agrumi ha prodotto non solo una perdita in termini economici, ma anche un impoverimento del paesaggio e una conseguente minore prevenzione dal punto di vista del dissesto. Negli ultimi decenni è evidente che il mutare delle condizioni climatiche ha accentuato il verificarsi di fenomeni di dissesto idrogeologico. Non possiamo, però, non constatare che l'abbandono delle zone marginali ha portato al verificarsi di fenomeni di dissesto laddove non si sono mai verificati quando l'attività agricola era presente. Per questo diventa strategico, per un Paese come il nostro, fare prevenzione attraverso il mantenimento delle attività in quei luoghi particolarmente fragili dal punto di vista ambientale. È un un paesaggio, quello italiano, così diversificato che necessita di un presidio costante e puntuale che solo l'attività agricola di qualità può garantire. E per questo diventa importante, anche in termini di prevenzione del dissesto idrogeologico, favorire e incentivare il ritorno all'agricoltura nelle zone marginali. In questo senso, ben vengano strumenti legislativi come quello in esame, che riconoscono agli agrumicoltori un ruolo a servizio della tutela ambientale indispensabile per certe aree del Paese. A mio parere, quindi, ben vengano dispositivi come questo, che sostengono sia il recupero degli agrumeti storici, sia i nuovi e vecchi imprenditori agricoli, che sono impegnati attraverso il lavoro a mantenere e preservare il paesaggio agrumicolo italiano.

Tuttavia, rimane immutata l'importanza e la necessità di concluderne l'approvazione, perché sappiamo quanto il settore agricolo versi in gravi difficoltà che persistono da molti, da troppi anni. Provengo da una Regione a vocazione vitivinicola, da un territorio che produce eccellenze e che ha saputo mettersi in discussione a partire dagli anni prediligendo a una produzione estensiva una produzione intensiva, quantitativamente ridotta e selezionata, che ha voluto guardare alla qualità della produzione anziché alla quantità. All'inizio poteva sembrare un'eresia rinunciare ai numeri della produzione, ma il tempo ha dato ragione a quella generazione di giovani imprenditori agricoli che hanno saputo compiere una scelta coraggiosa e, per molti versi, in antitesi al modo di pensare dei propri genitori e nonni. È l'esempio di una possibilità di scelta felice. Tuttavia, ci sono delle condizioni - il termine va inteso in senso letterale - che vanno oltre la volontà degli operatori e non permettono di scegliere, non permettono altre strade. Queste condizioni sono dettate dalla natura, dalla morfologia del territorio: per noi il costone carsico, che costeggia il mare sino a Trieste e ha caratteristiche morfologiche analoghe a quelle dei terreni destinati ad agrumeto, oggi oggetto di discussione. Anche in questo caso ci troviamo in una situazione in cui l'utilizzo dei macchinari è inibito dalla morfologia del terreno, il che comporta una lavorazione manuale. Anche in questo caso parliamo di piantumazioni intensive e non estensive. Anche in questo caso siamo in presenza di muri a secco che necessitano di continue manutenzioni. Anche in questo caso parliamo di zone soggette a rischio idrogeologico, che costituiscono un patrimonio storico nell'ambito della produzione di colture autoctone con modalità praticamente immutate nel tempo. Si tratta del territorio insulare delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico a rischio idrogeologico. Questo preambolo vuole significare che i provvedimenti contenuti nel disegno di legge odierno in particolare allo stanziamento di contributi a sostegno di quanti sfidano il tempo e le leggi della libera concorrenza dei mercati - sono indispensabili per salvaguardare sia il territorio, inteso come patrimonio, da un degrado e da un progressivo abbandono, sia le eccellenze agroalimentari che contraddistinguono, qui come altrove, il nostro Paese a livello globale. Con tutto il rispetto per la regolamentazione europea, che sappiamo indispensabile e alla quale abbiamo sottolineato nel provvedimento l'allineamento sulla base del principio contenuto nell'articolo 1 («Finalità»), non ci sono giustificazioni se per uniformare il mercato e le sue regole rischiamo di distruggere le peculiarità che contraddistinguono ciascun Paese della grande famiglia europea. Sono dunque indispensabili norme per la tutela, il recupero e la salvaguardia dei preziosi agrumeti caratteristici dei territori che sono di particolare pregio per il Paese. Si tratta dei terrazzamenti delle nostre fasce costiere, come la costiera amalfitana, il Gargano, le coste calabre e della Sicilia, il Garda, dove la coltivazione degli agrumeti rappresenta non solo una fondamentale fonte di reddito, ma anche un importante fattore di salvaguardia ambientale, conservativo dell'integrità dei territori ed equilibrio naturale costiero. Il provvedimento al nostro esame favorisce la conservazione dei paesaggi tradizionali e la tutela della biodiversità per valorizzare un prodotto dalle caratteristiche uniche. L'obiettivo dell'intervento legislativo è pertanto sostenere una delle coltivazioni caratteristiche del nostro territorio costiero e insulare nel Mediterraneo, rilanciando l'agrumicoltura italiana da anni in uno stato di profonda crisi; crisi determinata da costi di produzione insostenibili per la presenza di aziende di piccole dimensioni, poco raccordate tra di loro e con l'industria di trasformazione e la distribuzione; con strategie di promozione e commercializzazione obsolete, che non reggono più alla sempre maggiore concorrenza estera. L'asperità dei luoghi poco accessibili con mezzi meccanici - come ho già detto - determina il ricorso a un lavoro manuale che oggi è poco economico e faticoso sia per le colture che per il trasporto. Da ciò deriva l'abbandono da parte dei coltivatori, già evidenziato dalla collega che mi ha preceduto; coltivatori pochi e anziani che ancora praticano la cosiddetta agricoltura eroica, con il degrado del tessuto sociale e la perdita di un lavoro diventato con il tempo una parte fondamentale della cultura di quei territori, ma anche con la progressiva alterazione del paesaggio. sempre più vistosa la presenza di zone incolte e di danni all'assetto del territorio, privato della manutenzione degli agricoltori, sono sempre più visibili fenomeni di dissesto idrogeologico, per la perdita della funzione dei muretti a secco che i terrazzamenti svolgono nell'opera di contenimento sia delle acque che dei terreni. Come dicevo inizialmente per il costone carsico, va fermato il lento e inesorabile degrado e l'abbandono di quei territori, sostenendo chi opera per la salvaguardia di un inestimabile paesaggio rurale e di produzioni di qualità unica. Ecco perché voglio rivolgere un plauso ai parlamentari che hanno saputo concludere l'*iter* legislativo di un provvedimento molto atteso da tutti i produttori di agrumi, soprattutto da quelli più piccoli, che, con difficoltà e tanta fatica, hanno saputo resistere in questi anni, a costo di grandi sacrifici. A questi agricoltori va il merito, con riconoscenza, di mantenere vivo lo straordinario, spettacolare paesaggio costiero.

che il nostro Paese vede diffuse su tutto il territorio: si va dalle sponde del Lago di Garda fino alla costiera amalfitana, dalla Sicilia al Gargano.

Martina, mi dicono. Abbiamo perso il ricordo del volto. Ci resta scritto il nome da qualche parte sui giornali, ma certamente non ci dispiacerebbe poter godere della sua presenza, almeno per avere un confronto un po' più compiuto. In ogni caso, il ministro Martina - se è ancora Ministro

nel 2014, all'indomani dell'approvazione del provvedimento. Leggo testualmente: «"Recuperiamo e valorizziamo gli agrumeti caratteristici anche per difendere il territorio dal dissesto e la sua identità dall'abbandono". Lo affermano i parlamentari PD Nicodemo Oliverio e Colomba Mongiello, rispettivamente capogruppo e componente della Commissione agricoltura della Camera, commentando l'approvazione, in prima lettura, della legge sugli agrumeti caratteristici

o affacciati sul Garda garantiamo, per il tramite delle Regioni, un contributo finanziario di 4 milioni per il triennio 2014-2016 destinato a ripristinare, recuperare e salvaguardare gli agrumeti caratteristici

Non per nulla, nel provvedimento di legge sono state apportate dalla Commissione delle modifiche. Cito testualmente l'articolo 6 dove, al comma 2, è indicato che: «all'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016 Ovviamente, questo dice che il provvedimento, quando fu varato alla Camera, fu anche sostenuto con entusiasmo. Ma è altrettanto evidente che questo provvedimento e il contenuto, a parte che nel cuore dei firmatari e di chi l'ha sostenuto in Commissione,

e fare comparsate in televisione, non ha realmente coscienza e a cuore l'interesse delle coltivazioni del nostro territorio. Su questo c'è poco da fare e da dire. Il provvedimento è qui e sarà approvato certamente oggi, anche con delle sbavature e delle imprecisioni, perché prima il relatore mi ha confermato che non c'è intenzione di modificarlo - parole testuali del relatore, che invito eventualmente a smentire - altrimenti i tempi si dilungherebbero ulteriormente. Cari amici agricoltori, tenete conto che il provvedimento è qua fermo non perché l'opposizione non vuole approvarlo, ma perché la maggioranza non ha voluto portarlo in approvazione fino ad ora. Nel momento in cui, adesso, viene portato in approvazione, anche con delle difformità rispetto alla realtà, essendo passati due anni e mezzo, e viene chiuso velocemente, per non perdere altro tempo, diventa una ulteriore beffa, oltre al danno. Non è un modo serio di operare. Noi sosterremo il provvedimento. Lo sosteniamo perché siamo assolutamente convinti della necessità di tutelare le coltivazioni caratteristiche. anche se, con le premesse che ho appena fatto, ciò può avere un significato molto relativo - che non ci si può fermare a una singola coltivazione. Guai a limitare la visione

le altre coltivazioni tipiche che abbiamo opportunamente inserito nell'ordine del giorno G1.100, come le castagne.

un'agricoltura che va ben oltre i valori di mercato e che è radicata nel territorio proprio in quanto appartiene alla cultura di quelle terre, non limitandosi, ovviamente, a delle sollecitazioni.

di legiferare consenta anche ai singoli cittadini di poter avanzare petizioni che siano ricomprese e diventino addirittura il pilastro su cui si regge un intero provvedimento di legge. È un peccato che questa petizione si inserisca in un provvedimento che viene trascurato da due anni e mezzo. È significativo peraltro che ci sia stata questa sollecitazione, che nasce quindi non esclusivamente da interessi di categoria, ma anche da una considerazione che ripeto e ripeterò ancora in dichiarazione di voto: la nostra è un'agricoltura che ha delle peculiarità, che devono essere difese.

ma è un territorio che nelle sue bellezze, come lo conosciamo, deriva da una straordinaria commistione tra aspetti naturali e aspetti antropici, con le persone che, con il loro lavoro e con l'agricoltura, hanno modificato e modellato il territorio, fino a renderlo nell'unicità in cui oggi lo conosciamo e che ci viene invidiata da tutto il mondo. Proseguiamo con questo provvedimento, pur non essendo soddisfatti - lo ripeto - perché abbiamo già intuito che anche gli emendamenti che chiedono maggiori stanziamenti saranno respinti. Insisteremo in ogni opportunità di legge perché i finanziamenti inseriti in questo provvedimento siano ulteriormente estesi e affinché le stesse regole che vengono messe a tutela degli agrumeti caratteristici siano estese anche alle altre coltivazioni cui ho poc'anzi accennato.

Si tratta di un provvedimento che tende a salvaguardare e a valorizzare alcuni areali caratteristici coltivati storicamente ad agrumi. Si tratta principalmente di alcune zone ubicate nella riviera ionica della Sicilia, nella riviera ionica e tirrenica della Calabria, nella penisola sorrentina, nella costiera amalfitana e nelle isole del Golfo di Napoli, nel Gargano e intorno al lago di Garda. La storia dell'agrumicoltura tradizionale italiana affonda le sue radici in epoca romana, per raggiungere il massimo di espansione economica intorno alla metà del Settecento; le aree di produzione si svilupparono prevalentemente intorno al mare, per la presenza di un clima temperato e la possibilità di sopperire alla mancanza di piogge con interventi di irrigazione. In epoca contemporanea tali zone hanno subito un arretramento dal punto di vista commerciale, anche a causa dei crescenti costi di produzione, delle ridotte dimensioni delle aziende e delle difficoltà di raccordo con la grande distribuzione. Servono pertanto degli interventi *ad hoc* per garantire la tutela di produzioni tipiche e, di conseguenza, il sostegno ad aziende che non possono competere, per costi e produzione, con le sfide della globalizzazione. Anche queste azioni permettono la tutela della biodiversità agraria, fondamentale per tutelare le eccellenze del *made in Italy* e delle coltivazioni del bacino del Mediterraneo. Oltretutto, i soggetti interessati dagli interventi svolgono un importante presidio del territorio in zone territoriali a forte rischio di spopolamento e di dissesto idrogeologico. Pertanto, il testo licenziato dopo un lavoro certosino da parte della Commissione agricoltura del Senato ha come scopo il ripristino, il recupero, oltre che la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, dove per agrumeti caratteristici si intendono quelli aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale e che sono situati in quelle aree particolarmente vocate alla produzione di agrumi e nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche rendono il prodotto unico nel suo genere proprio perché strettamente legato al territorio. Si prevedono specifici interventi sia per il recupero e la salvaguardia degli agrumeti caratteristici sia per gli interventi di ripristino di quelli abbandonati. Per tali interventi si prevede uno stanziamento di 3 milioni per il 2017, da ripartire fra i territori interessati. Viene precisato, al riguardo, che i contributi sono concessi in via prioritaria per lo sviluppo di tecniche di allevamento tradizionale e per l'agricoltura integrata e biologica, oltre che per interventi che facilitino in modo prioritario l'utilizzo di tecniche sostenibili connesse all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e valorizzino la tradizione delle entità locali. Il provvedimento prevede, infine, una serie di controlli e le sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nel testo. Nello specifico, si prevede che, nel caso in cui gli interventi siano realizzati in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella domanda, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato; il soggetto responsabile è altresì escluso dalla possibilità di ottenere in futuro i contributi. Nel caso in cui, invece, gli interventi indicati nella domanda non vengano realizzati affatto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Viene, anche in tal caso, confermata l'esclusione dalla possibilità di partecipare all'erogazione di ulteriori contributi. Questo testo rappresenta un'evoluzione in chiave migliorativa del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento qualche anno fa. Adesso, dopo l'approvazione unanime da parte della Commissione agricoltura, auspico una rapida approvazione del provvedimento alla Camera in via definitiva, prima della fine della legislatura. Spetterà poi al Governo, d'intesa con le Regioni, individuare le aree di intervento da tutelare. Salvo inciampi, finalmente arriverà il giusto riconoscimento legislativo a questo patrimonio, più storico e ambientale che semplicemente agricolo. Saranno quindi preservate da una legge, ad esempio, le limonaie, manufatti architettonici unici al mondo che fin dal XV secolo modificarono a finalità produttive il paesaggio della sponda bresciana del lago da Salò fino a Limone. in discussione riconosce il legame degli agrumi con il territorio d'origine, il fatto d'esserne un elemento di caratterizzazione e quindi anche di tutela e giusta valorizzazione. Questo provvedimento è l'ennesimo passo per la valorizzazione delle eccellenze italiche.

non può non richiamare all'attenzione e alla memoria di quest'Assemblea alcuni riferimenti, se volete di natura letteraria, perché gli stessi possono essere presi ad esempio esempio e come archetipo dell'importanza del paesaggio così come venutosi a formare per azione naturale e per virtuosa azione umana nei secoli. Il riferimento è quello abbastanza conosciuto al romanzo di formazione di Wolfgang Goethe «Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister» alla frase più o meno nota: «Conosci tu il Paese dove fioriscono i limoni? Brillano tra le foglie cupe le arance d'oro». Penso che in queste due righe

Ebbene, non si può non essere d'accordo con lo spirito e i contenuti del disegno di legge. Non si può pensare che

la necessità di tutelare le coltivazioni caratteristiche di agrumeti anche ad altri tipi di *cultivar*, ad altre colture, direi ad altre varietà di ortofrutta, le stesse che poi hanno contribuito a dare forma e sostanza ad alcuni angoli caratteristici, suggestivi e affascinanti della nostra Penisola. indicate nel provvedimento, come giustamente il lago di Garda, vorrei aggiungere una peculiarità che riguarda il Gargano e la fascia ionica pugliese e lucana, così fortemente contrassegnati dalla presenza di queste colture estensive e L'auspicio è quello, appunto, di prendere in considerazione anche questi luoghi dimenticati del nostro Paese, tutto vantaggio della biodiversità e della biotipicità che finalmente tornano a essere principi cardine delle produzioni agricole e quindi anche di quelle eccellenze del cosiddetto *made in Italy* a cui il disegno di legge in esame vuole dare un contributo di valorizzazione.

Oggi c'è già, è condivisa e abbastanza sancita l'idea in agricoltura, nel settore vitivinicolo, dei cosiddetti vigneti storici, quelli molto peculiari e in cui esiste la necessità di salvaguardare lo spirito tradizionale e antico. Sono vigneti cosiddetti eroici, perché il concetto è esteso alla qualità e alla quantità di tempo che gli operatori dedicano affinché queste *enclave* del nostro paesaggio resistano, resistano da tutti i punti di vista, compreso quello del Con questo spirito, siamo abbastanza favorevoli affinché il provvedimento venga quanto prima

un disegno di legge che proviene, a sua volta, da un testo unificato approvato alla Camera, frutto di un lavoro istruttorio che si è originato nelle precedenti legislature e che poi è stato ripreso in quella attuale attraverso la presentazione di numerose proposte in materia. Un'opera di copia e incolla, tramandata negli anni, a cui si è accostato lo svolgimento di un ciclo di audizioni per disporre di un quadro conoscitivo completo. Per molto tempo, perciò, questo Atto Senato 1641, recante disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, ci ha fatto compagnia tra una seduta di Commissione e l'altra, anche se, per la verità, sono dovuti passare molti mesi (da ottobre del 2015 al febbraio del 2017) perché si passasse dalla mera illustrazione degli emendamenti alla votazione vera e propria, sempre in 9a Commissione. Fatte queste considerazioni iniziali, il quadro deve essere arricchito dalla situazione attuale, una situazione davvero poco confortante, con un *export* di agrumi ridotto all'osso ed una importazione che stona con la vocazione ed il clima del nostro territorio. Sappiamo, secondo gli ultimi dati disponibili, che tra il 2010 ed il 2015, l'Italia ha importato ben 2,3 milioni di tonnellate di agrumi con una spesa di quasi due milioni di euro. Si tratta di una media di 390.000 tonnellate di prodotto importato ogni anno, pari ad una somma, sempre per anno, di 290 milioni

il 1999 e il 2016, i Paesi dell'Unione europea hanno importato - sempre dall'Africa australe - oltre 10 milioni di tonnellate di agrumi, di cui la prevalenza sono proprio arance. Questa incessante tendenza ha giocato un brutto colpo non solo alle colture ordinarie di agrumi presenti in Italia, ma soprattutto a quelle caratteristiche, la cui tipicità e tradizionalità si è persa pian piano. In un contesto globale sempre più competitivo, la difesa del territorio e la conservazione dei paesaggi tradizionali hanno, perciò, subito un forte attacco. Purtroppo, infatti, non bastano delle buone e, in alcuni casi, ottimali caratteristiche orogeografiche per determinare la fortuna di un territorio e dei suoi prodotti agrumicoli. Occorrono anche una costante cura, un'organizzazione razionale della filiera, infrastrutture logistiche efficienti e la presenza di enti ed organismi che siano in grado di promuovere la diffusione, attraverso il commercio capillare, dei frutti raccolti. Le indagini strutturali parlano di un calo del 22 per cento - dal 2010 al 2013 - delle aziende agricole operanti nel settore, che ha letteralmente condannato i tantissimi coltivatori diretti e piccoli imprenditori che avevano investito nel campo, puntando alla valorizzazione del patrimonio rurale. Ora, visto che il testo ha cambiato formulazione rispetto alla lettura alla Camera, è evidente che verrà esaminato in una successiva terza lettura. Evenienza, questa, che fa cadere nel vuoto l'esigenza di dare una pronta legislazione alla materia. Ci chiediamo, quindi, che senso abbia questa pratica, che svilisce i lavori parlamentari e che li esautora. Detto questo, ci auguriamo che la trattazione di questo disegno di legge in Aula non rappresenti uno dei tantissimi tentativi dilatori attuati da questo Governo. Sarebbe l'ennesima presa in giro nei confronti di milioni di italiani che non vedono l'ora di votare, per dimenticare, una volta per tutte, questo triste e finale scampolo di legislatura senza capo né coda.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo esaminando reca norme per il recupero e la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare valore paesaggistico, nell'ambito delle più ampie finalità, di competenza statale, relative alla tutela ambientale, alla difesa del territorio e del suolo, alla conservazione dei paesaggi tradizionali e alla valorizzazione della biodiversità agraria. Come dispone l'articolo 1, si prevedono interventi di ripristino, valorizzazione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici, ovvero quelli ubicati nelle aree vocate alla loro coltivazione, dotate di particolari condizioni ambientali e climatiche, che conferiscono al prodotto caratteristiche uniche e strettamente connesse alle peculiarità del territorio di provenienza. Gli obiettivi della tutela e della valorizzazione della biodiversità agraria e la salvaguardia di alcune aree caratteristiche coltivate storicamente ad agrumeti riguardano numerose aree della nostra Penisola, compresa la Sicilia orientale e Sud-orientale. Le norme al nostro esame, dunque, incidono in via prioritaria sull'aspetto ambientale-paesaggistico ma non è da trascurare, oltre al sostegno economico previsto dal fondo all'articolo 6 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, l'aspetto relativo alla promozione indiretta del benessere fisico legato a una più sana alimentazione. Infatti, il rafforzamento al sostegno della produzione di agrumi, come previsto anche dalle norme sulle attività dei consorzi di tutela, si pone anche l'obiettivo di migliorare la resa produttiva e far rivivere agrumeti posti in zone impervie o abbandonate, con l'obiettivo di riavvicinare le comunità locali al consumo di prodotti tipici del territorio. Questo può avere effetti diretti sul consumo di agrumi nel nostro Paese, peraltro in ragione dei numeri che riguardano il settore, aiutando ad assumere stili di vita più corretti, invitandoci a scegliere prodotti salutari, quelli a chilometri zero. Penso soprattutto ai ragazzi, ma anche a noi adulti, che troppo spesso ci facciamo prendere dall'utilizzo di bevande certamente non innocue, molto zuccherate, che non aiutano a mantenere il nostro benessere. Perché non scegliere, invece,

con 130.000 ettari di superfici coltivate: qui, come in altre zone d'Italia, sono coltivati quei prodotti di qualità, dall'elevato valore nutrizionale, che rappresentano un simbolo caratteristico dell'isola. Considerando gli aspetti storici che legano gli agrumi a molte aree dell'Italia meridionale e insulare, certamente la Sicilia risulta essere tra quelle più strettamente correlate alla produzione agrumicola, anche grazie all'utilizzo storicamente compiuto delle piante di agrumi in funzione di abbellimento di giardini e palazzi. Gli agrumi, così come le palme, fanno parte del nostro paesaggio, come se fossero dei monumenti viventi,

(e non solo: pensiamo, ad esempio, alla zona del lago di Garda), è per natura legata alle produzioni agrumicole grazie alla presenza di un clima temperato e piuttosto mite anche d'inverno. In generale, l'agrumicoltura, nel nostro Paese, ha avuto crescita progressiva che spesso si è modellata intrecciandosi con la storia dei territori dove veniva praticata: l'arancia rossa di Sicilia è intimamente legata, anche nell'immaginario collettivo, alla stessa cultura di alcune Province sicule e certamente è legata ai paesaggi e alle tradizioni delle comunità locali. Pensiamo alle varietà Tarocco, Moro e Sanguinello, che sono note in tutti i mercati nazionali e rappresentano un fiore all'occhiello per le Province di Ragusa, di Siracusa e di Catania. È fondamentale, quindi, prevedere interventi che ripristino e valorizzino condizioni commerciali, sociali e culturali relative alla produzione agrumicola, che sono mutate nel corso del tempo, a volte facendo perdere, nelle aree interessate, importanza a quella fonte di benessere che gli agrumi rappresentano per l'intero nostro Paese e, in particolare, per il Mezzogiorno. importantissimo sostenere la rivitalizzazione di zone abbandonate, per via di condizioni di coltivabilità che sono divenute sempre più difficoltose e onerose, poiché con questi interventi si possono ottenere benefici, come ben sottolineato nel a livello sia di tutela del paesaggio, che di salvaguardia dell'ambiente. Inoltre, si contribuisce a ridare slancio a tradizioni che per lungo tempo sono state punto di forza di una cultura nazionale fondata, *in primis* al Sud, sulla coltivazione della terra, aiutando concretamente quanti conducono un agrumeto e versano in condizioni di difficoltà. Si pensi, per esempio, agli ostacoli che può incontrare un imprenditore agricolo o un coltivatore diretto

Mi piace sottolineare l'aspetto della norma in esame che incoraggia sicuramente sempre più la presenza dei giovani che stanno tornando a prendersi cura della terra e dell'agricoltura, stigmatizzando sempre di più l'intreccio tra tradizione, storia, innovazione e quel valore etico e sociale che riveste l'agricoltura stessa. Abbiamo detto che intervenire per salvaguardare e ripristinare dove necessario, tali produzioni ha un rilievo particolare ai fini della tutela paesaggistica. Il degrado dei terrazzamenti e l'abbandono di luoghi impervi comportano l'impoverimento dei suoli, con i conseguenti rischi legati, come già detto, al divallamento dei relativi pendii, che possono causare danni piuttosto seri dal punto di vista idrogeologico. L'intervento L'intervento legislativo, dunque, si pone in linea di continuità con quanto stabilito nella Convenzione del 2000 del Consiglio d'Europa per la definizione di regole comuni per la protezione, la pianificazione e la gestione dei paesaggi nel diritto internazionale. Essa afferma la centralità della tutela paesaggistica quale componente indispensabile delle strategie di gestione del territorio di competenza degli Stati aderenti. La disciplina degli interventi, demandati dal provvedimento alla competenza regionale, prevede la concreta individuazione dei territori in cui sono situati gli agrumeti caratteristici e la definizione di criteri e tipologie per cui è concesso il contributo pubblico statale. In quest'ambito, vale rammentare come gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi debbano prioritariamente rispettare tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e debbano essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati alla protezione delle caratteristiche di tipicità delle comunità locali. In questo modo, il legame tra la tutela del paesaggio e dell'ambiente si fonde con la valorizzazione della biodiversità agraria, contribuendo a raggiungere gli scopi prefissati dalla legge. Infine, un ultimo rilievo cui accennare riguarda gli effetti indiretti quale occasione di impulso e incoraggiamento finanziario per il supporto alla filiera agroalimentare, anche in ragione del peso relativo (circa il 7 per cento) che essa riveste nell'*export* nazionale. Nonostante *trend* recenti in rialzo, di fatti, la bilancia commerciale del settore è nel complesso negativa a causa del *deficit* di produzioni agricole rispetto alle necessità dell'industria alimentare e al carico che

intervenendo sui meccanismi che riguardano la produzione e la distribuzione di prodotti tipici dei nostri territori costieri. Certamente il trasporto di prodotti e merci su gomma, che è di gran lunga la modalità più utilizzata nel nostro Paese, non contribuisce a ridurre i costi sostenuti dalle imprese agricole, abbassando in via generale l'efficienza della filiera agroalimentare, che risente delle inefficienze del sistema Paese. Per questo motivo, occorre attuare strategie di ampio respiro che, ripartendo da una rinnovata centralità per la terra e per i suoi prodotti, si pongano l'intento di salvaguardare, tutelare e rendere sempre più competitive le produzioni locali, oltre a quello della tutela paesaggistico-ambientale, riconoscendo il valore nazionale di un inestimabile paesaggio formato da un intreccio secolare di natura e cultura.

Questo vale per la Sicilia e per tutte le altre zone coinvolte: pensiamo al Garda, al Gargano o alla Calabria. Tutte queste zone, di cui abbiamo parlato nel provvedimento

Signora Presidente, il mio sarà un intervento molto breve. Vorrei soprattutto ricordare

e, tra un balletto e l'altro, del provvedimento non si è più parlato, se non qualche mese fa.

territorio e penso di poter dare, come ho fatto anche in Commissione, il piccolo contributo di chi si occupa quotidianamente di queste attività.

perché ci sono tanti agrumeti cosiddetti terrazzati, che stanno cioè sulle terrazze, che poter coltivare è ormai diventata una tragedia, perché i costi sono enormemente maggiori degli eventuali ricavi.

il collaudo del MOSE è costato alle tasche dei cittadini 19 milioni di euro.

possa corrispondere al sostegno a un'attività così importante e significativa qual è l'agrumicoltura italiana. Io penso di no. Certo, so che non è possibile fare nulla in questi momenti e anche io voterò convintamente il provvedimento nonostante queste sottolineature.

una più generale esigenza di mettere in sicurezza colture e culture. Mi riferisco in questo caso a quella degli agrumeti, che caratterizzano il nostro paesaggio, il nostro territorio e che sono il testimone che dovremmo consegnare alle nuove generazioni.

è troppo difficile immaginare il disegno completo, ma rappresenta un tassello di un mosaico più ampio che dovremo continuare a costruire, non attraverso normative nazionali, ma con un nostro impegno più significativo nel quadro europeo. Da europeista convinto, penso che ci ritroviamo nella necessità di interpretare strumenti normativi nazionali per difendere, recuperare e valorizzare le nostre identità culturali e paesaggistiche, perché per troppo tempo abbiamo abbracciato un'idea di Europa che ha tentato di standardizzarci non dandoci la possibilità di mettere in evidenza le particolarità dei singoli territori. Credo che dovremmo impegnarci su anche in forza di quanto sta accadendo negli ultimi anni: queste nostre culture e colture caratteristiche sono sempre più minacciate da emergenze fitosanitarie, frutto di una globalizzazione senza regole che l'Unione europea non ha saputo dirigere con il piglio di chi doveva invece determinare condizioni di tutela. Il provvedimento di oggi quindi va bene, anche se è un provvedimento che non può essere esaustivo né per gli agrumeti né per le nostre peculiarità produttive, ma pensiamo a cosa sono per noi gli ulivi secolari, cosa sono le viti, cosa è tutto quel patrimonio paesaggistico che abbiamo il compito di valorizzare. Ben venga allora questo provvedimento, anch'io lo ho condiviso in Commissione e lo condivido qui in Assemblea, ma solo se esso rappresenta il viatico di un nuovo impegno che andiamo ad assumere in un'Europa che vorremmo ci accompagnasse in questi processi di recupero delle nostre identità. Un Paese come il nostro, riconosciuto in tutto il mondo come Paese a maggior significato nelle produzioni primarie e nelle specificità paesaggistiche territoriali, ha la necessità di ricominciare, investendo sulla propria identità, sulla propria storia, sui testimoni che ci vengono consegnati da generazioni di agricoltori. proposito mi viene facile dire che un Paese che non investe nella valorizzazione del proprio passato è un Paese che non ha prospettiva.

che di questi provvedimenti in futuro non ci sia più bisogno, perché avremo avuto la possibilità di incidere su politiche europee che ci consentono di salvaguardare e valorizzare le nostre identità e non di difenderle dalle imitazioni. Finché l'Europa consentirà di avere un'indicazione geografica protetta

avremo anche la forza di varare provvedimenti di valorizzazione come questo, ma saremo destinati a perdere, perché la nostra battaglia dobbiamo consumarla su quel fronte e non attraverso singoli interventi normativi, peraltro con risorse finanziarie sempre troppo scarse per vincere una sfida che potremmo vincere invece con maggiore agilità.

operare in sede legislativa su provvedimenti di natura agricola. Mai come in questa legislatura sono stati approvati provvedimenti di ampia portata nell'ambito dell'agricoltura che molto hanno avuto a che fare con la materia specifica. Siamo intervenuti a fronte di crisi di settore, ma anche per la riorganizzazione intera delle filiere. Basti pensare al progetto Campolibero all'ultimo importante lavoro che è stato il collegato agricoltura. Questo è, a mio avviso, particolarmente importante

Questo elemento, che spesso avevamo semplicemente evocato nei decenni passati, è diventato in realtà una scelta strategico-politica di questi ultimi anni. Il nostro Governo, anche attraverso la scelta della tracciabilità dei prodotti, in ultimo il latte e i latticini, ma anche il grano duro e il riso,

di cultura tradizionale, di cultura agricola, ma anche patrimonio ambientale e paesaggistico. È vero: il provvedimento non è esaustivo, ma va nella giusta direzione. È un provvedimento - non dimentichiamolo mai, colleghi che interpreta quanto il Parlamento ha scelto per l'ambito agricolo, e cioè che il nostro fosse il Ministero «delle politiche agricole». Abbiamo poi gli strumenti adatti al finanziamento, abbiamo investimenti territoriali fatti dalle nostre Regioni, che naturalmente devono essere indirizzati politicamente, come facciamo con queste ma che esistono e sono cospicui e possono interagire per andare a riempire di senso e contenuto il provvedimento stesso. Noi abbiamo collocato alcune risorse, altre potranno aggiungersi, senza dubbio a livello nazionale ma ancora più, ribadisco, a livello territoriale.

per i nostri territori, e anzi consideriamo fondamentale il compito di salvaguardia di questo come di tanti altri specifici settori agricoli che sono vera rappresentazione della cultura italiana; non di una cultura minore ma di una grande cultura che fa grande l'Italia nel mondo. Concludo ringraziando tutti i colleghi che si sono adoperati in questi mesi passati per accelerare il percorso. Ringrazio il senatore Scoma, relatore del disegno di legge, e quanti in Commissione hanno voluto fortemente il provvedimento

Avverto che la Presidenza dichiara inammissibile l'emendamento 2.4 in quanto diretto a rendere vincolante il parere che le Commissioni permanenti di entrambe le Camere dovranno esprimere in relazione

La previsione di un parere parlamentare di natura vincolante in relazione ad un potere normativo, legislativo delegato o regolamentare attribuito al Governo si pone, infatti, in contrasto con il riparto di competenze tra organi dello Stato stabilito direttamente dalla Costituzione sul quale il legislatore ordinario non può incidere. Il carattere vincolante di un parere parlamentare, inoltre, non appare conforme ai canoni di ragionevolezza e di correttezza istituzionale in quanto i pareri resi da ciascuna Camera potrebbero potenzialmente esprimersi in senso difforme, rendendo conseguentemente impossibile l'adozione della normativa delegata.

a valutare l'adozione di disposizioni legislative, similari a quelle previste nel disegno di legge all'esame, per tutte quelle produzioni agricole, quali ad esempio la vite di montagna, i castagneti, le erbacee minori, quali le piante officinali, nonché tutti i prodotti spontanei di montagna e del territorio,

rispondenti alle caratteristiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge.

L'emendamento 4.102 vuole inserire all'interno della priorità anche i piccoli imprenditori agricoli e le imprese a conduzione familiare.

Signora Presidente, l'articolo 7 è particolarmente importante in quanto stabilisce le procedure per l'assegnazione dei contributi.

Il Vice Ministro prima faceva riferimento al PSR e ai fondi europei che vengono percepiti. Voglio ricordare che nel passato settennio abbiamo perso 1,8 miliardi del PSR e sono in fase di contrattazione 2,2 miliardi per per quel che riguarda i fondi europei. Occorre quindi usare la massima trasparenza sulla destinazione dei soldi pubblici. Credo che questa sia la miglior forma di controllo, perché quando il vicino di casa si accorge che l'altro percepisce somme di denaro non dovute la cosa risulta molto interessante.

come già fatto precedentemente, la responsabilità di avere tardato di due anni e mezzo l'approvazione di un provvedimento su cui si è trovata una così ampia convergenza nell'Assemblea del Senato.

preservando la coltivazione degli agrumeti tradizionali e soprattutto la cultura che è legata alla coltura degli agrumi. Lo stesso sia fatto per le castagne e per le altre coltivazioni tipiche. Se ci saranno anche i fondi a disposizione ci dichiareremo soddisfatti ed esprimeremo un ulteriore plauso al Governo; se questo non avverrà saremo i più grandi castigatori nei confronti del Governo, perché non si possono illudere i cittadini con leggi che poi non sono finanziate.

poche parole per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo, Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista, al provvedimento oggi al nostro esame. Si tratta di un voto favorevole, perché il provvedimento contiene norme per il recupero e la salvaguardia degli agrumeti caratteristici che, come specificato dal comma 2 dell'articolo 1, sono quelli di particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarità del territorio di origine. L'obiettivo del provvedimento, quindi, è quello della più ampia finalità di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo, di conservazione dei paesaggi tradizionali e di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria. Molti in discussione generale hanno citato Goethe e allora, se il nostro Paese è quello dove «fioriscono i limoni e ardono le arance dorate fra il fogliame scuro», noi dobbiamo proteggere tutto questo, curarlo, salvaguardarlo e se necessario ripristinarlo. È previsto un ampio coinvolgimento delle Regioni nell'attuazione della legge; è richiesta l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul decreto ministeriale che deve individuare i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici; nello stesso decreto vanno definiti i criteri e le tipologie degli interventi previsti ammessi ai contributi e deve essere determinata la misura dei contributi erogabili. La Regione interessata definisce l'ammontare delle risorse da destinare ai contributi, stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari, oltre che all'erogazione dei contributi stessi, che sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il provvedimento mette a disposizione per l'anno 2017 un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro. Questo impegna tutti a fare presto, in modo da non vanificare il finanziamento, come purtroppo è successo con quello previsto per il 2016, che il lungo *iter* del provvedimento non ha permesso di utilizzare proficuamente. *(Applausi

un'importante convergenza. La Commissione ha approvato il provvedimento all'unanimità e siamo quindi soddisfatti di poter esaminare e - spero - approvare il testo definitivo in tempi finalmente ravvicinati. Ringrazio quindi tutti i presentatori, il relatore Scoma e il vice ministro Olivero per l'importante lavoro svolto insieme ai componenti della Commissione agricoltura

individuano come beneficiari prioritari i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli locali, con un occhio di riguardo al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati che con il provvedimento in esame speriamo possano essere salvati e recuperati Il provvedimento in esame interessa dunque tutta Italia e, per quanto riguarda la mia esperienza diretta, anche le storiche limonaie del Garda, potendo contribuire alla loro salvaguardia e al mantenimento di una specificità come elemento di valore economico, paesaggistico e anche culturale del territorio. La presenza degli agrumeti e delle loro coltivazioni caratteristiche concorre innanzitutto al mantenimento della biodiversità e della tipicità vegetazionale, ma anche all'attrattività turistica del nostro Paese. Credo che tutti in quest'Aula abbiano in mente le bellissime limonaie della costiera del Garda, che, con le caratteristiche strutture di protezione realizzate molti decenni fa dai contadini, emergono dalla flora mediterranea, connotando in maniera inconfondibile lo splendido paesaggio del lago. Purtroppo alcune limonaie sono andate distrutte, altre sono state recuperate in interventi edilizi che ne hanno comunque salvato la particolarità architettonica, altre sono ancora coltivate e altre sono state recuperate in questi ultimi anni, anche se purtroppo, a seguito della costruzione della galleria Adige-Garda,

Ricordo che sono circa 170.000 gli ettari di agrumeti in Italia, in prevalenza in Sicilia e Calabria, ma anche in altre Regioni. Si tratta, dunque, di un patrimonio che va difeso e rilanciato perché ha grande potenzialità. Arance, limoni, mandarini e mandaranci italiani sono prodotti di altissima qualità, controllatissimi dal punto di vista fitosanitario e che si prestano anche a trasformazioni industriali che non si limitano a succhi e marmellate, in quanto, grazie a tecnologie innovative, si può arrivare a sfruttarne in maniera virtuosa anche gli scarti. In questo settore dai grandi numeri è perciò necessaria una strategia complessiva di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'agrumicoltura italiana e di tutta la sua filiera: produzione, commercializzazione e trasformazione. L'agrumicoltura nel corso dei secoli è stata caratterizzata da una progressiva crescita, tale da modellare e condizionare la società, il territorio e l'ambiente dove veniva praticata, diventando, per estesi comprensori, parte integrante con il territorio e con le tradizioni popolari. Questo settore, che rappresentava una fonte di benessere nei decenni passati, ha subito dagli anni Sessanta in poi una sempre più accentuata perdita d'importanza a causa delle mutate condizioni commerciali, sociali e culturali, da ricondurre a diversi fattori, tra cui i crescenti costi di produzione, le ridotte dimensioni delle aziende e la concorrenza estera sempre più forte e aggressiva. Il risultato di tale processo si è concretato in uno stato di crisi certamente aggravatosi negli ultimi decenni, che ha provocato molto spesso l'abbandono di quelle aree in cui le condizioni di coltivabilità erano più difficili e onerose, con conseguente impatto negativo sia a livello paesaggistico che di salvaguardia del territorio e con riflessi gravi, anche con riferimento all'abbandono di quelle tradizioni che sono state un punto di forza della cultura e dell'identità italiana.

la Basilicata con il 4,7 per cento e la Campania con il 2 per cento e anche altre Regioni, tra cui mi sia permesso di ricordare, sia pure in termini minori, la stessa Lombardia, sulle costiere gardesane. Negli ultimi due decenni il comparto agrumicolo nazionale ha subito notevoli cambiamenti in termini sia di offerta sia di domanda, ricalcando quanto registrato anche in altri settori produttivi. Essi hanno riguardato l'aumento dei costi del lavoro e dei mezzi tecnici, l'inasprimento delle politiche fiscali e previdenziali, la riduzione dei prezzi alla produzione e lo smantellamento delle politiche comunitarie di tutela e di sostegno del reddito degli agrumicoltori, che hanno determinato una situazione critica e, a volte, gravemente critica. A livello della produzione questo stato si è accentuato soprattutto negli ultimi cinque-dieci con forti squilibri fra costi e ricavi, che hanno portato alla conseguente minore attenzione nei confronti della coltura, determinando, in alcuni casi, persino l'abbandono dei campi, con effetti negativi sulle produzioni, sui redditi e sull'occupazione dell'intera filiera agrumicola nazionale. Gli operatori del comparto hanno comunque molto spesso reagito, ad esempio attraverso l'introduzione di un'ampia gamma di innovazioni tecniche, da quelle specificatamente agronomiche, basate su modalità di conduzione degli impianti diverse dal passato per irrigazione e gestione del suolo, all'adozione di protocolli nuovi per le produzioni biologiche. Come spesso accade in frutticoltura, l'innovazione è immediatamente intesa e percepita quando si parla di nuove varietà e portinnesti, che tendono a soddisfare l'adattamento del prodotto alla domanda dei mercati e così spesso è avvenuto. Appare di significativo rilievo ricordare che il provvedimento in esame è il frutto di un lungo lavoro istruttorio, che trae origine - è vero - dalle precedenti legislature, con particolare richiamo alle iniziative della legislatura scorsa, a dimostrazione di quanto la rilevanza della problematica e l'esigenza di intervento siano avvertite dalle diverse forze in sede politica e parlamentare. Il provvedimento ha trovato in questa legislatura una particolare attenzione, specialmente nella Commissione che ho l'onore di presiedere. Esso prevede anche la concessione di un contributo a copertura parziale delle spese per il recupero e la salvaguardia degli agrumeti, e un contributo unico a copertura parziale delle spese per sostenere il ripristino degli agrumeti abbandonati. Per tali interventi si prevede uno stanziamento di 3 milioni per l'anno 2017, da ripartire fra i territori interessati. Viene precisato, al riguardo, che i contributi sono concessi in via prioritaria per lo sviluppo di tecniche di allevamento tradizionale e per l'agricoltura integrata e biologica, oltre che per interventi che facilitino in modo prioritario l'utilizzo di tecniche sostenibili connesse all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e valorizzino la tradizione delle entità locali.

voglio anche sottolineare l'approvazione unanime da parte della Commissione agricoltura e auspicare non solo un vasto voto a favore del provvedimento da parte di questa ma anche un interesse immediato della Camera dei deputati affinché il varo definitivo della legge possa avvenire in termini altrettanto rapidi. Ricordo, infine, che il provvedimento riconosce il legame degli agrumi con il territorio d'origine, il fatto di esserne un elemento di caratterizzazione e, quindi, anche di tutela e giusta valorizzazione.

molto d'accordo con un disegno di legge che ha come obiettivo fondamentale la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Dispiace che il provvedimento arrivi ad approvazione dopo due anni e mezzo.

Sono circa 130.000 gli ettari dedicati alla coltivazione degli agrumi e questi hanno formato il paesaggio di moltissime zone; sono un elemento certamente d'identità. Vorrei ricordare a me stessa e a questa

i sistemi agricoli che hanno caratterizzato in modo particolare la storia di alcuni territori e dei paesaggi contribuendo a quel lavoro importante che è il Catalogo nazionale dei paesaggi rurali

delle caratteristiche tradizionali del paesaggio agrario, ma dobbiamo anche renderci conto che vi è una crisi dell'intera filiera sia della coltivazione, che della trasformazione. I dati di mercato diffusi anche recentemente dall'Ismea indicano che vi è una grave crisi di redditività

con punte al ribasso dei prezzi, registrate nel corso della campagna 2015-2016, fino a sette centesimi al chilo.

in particolare dal Nord Africa, e quello dei ritardi strutturali di tutto il comparto in termini di organizzazione dei produttori, di infrastrutture per il trasporto e di *marketing*. Si sta quindi sempre più aggravando una situazione che - ahimè - rischia

degli indirizzi per un piano di settore per l'agrumicoltura, con degli idonei finanziamenti per il prossimo triennio,

all'integrazione con il comparto della trasformazione e quindi a fare in modo di sostenere l'anello più debole della catena, cioè i produttori agricoli,

Signor Presidente, se in questi giorni le capiterà di venire in Sicilia e di atterrare all'aeroporto di Catania o anche di Palermo,

Se poi si cammina per le strade che attraversano questi aranceti, si sente un bellissimo odore: un profumo

che hanno imparato a coltivare quest'oro. Intere generazioni che, giorno dopo giorno, nel corso di centinaia di anni hanno affinato una coltivazione straordinaria. Quando si parla di peculiarità, di caratteristiche tipiche di un prodotto, vorrei ricordare a tutti in questa Aula, per quanti non lo sanno - so che molti non ne sono a conoscenza l'arancia rossa siciliana è un *unicum* al mondo; lo è perché quella colorazione rossa straordinaria è tale perché solo lì si forma.

peculiare dell'arancia rossa siciliana. Alle antocianine è legata la straordinaria capacità agroalimentare e organolettica dell'arancia,

affidare il proprio benessere e il benessere dei propri figli. Tutto questo è stato messo in crisi da una serie di meccanismi, soprattutto da quella globalizzazione che ha portato a introdurre nel mercato arance di altre parti del mondo (dove

Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo provvedimento. Purtuttavia io vorrei chiarire, soprattutto a me stesso, alcuni interrogativi: stiamo parlando della politica agrumicola nazionale o stiamo parlando di agrumeti caratteristici? Perché se parliamo della politica agrumicola nazionale, ridursi a un fondo di tre milioni per il 2017, ricavato all'interno degli stessi fondi del Ministero delle politiche agricole, mi sembra cosa ben riduttiva: anzi, preoccupante. Come sempre, poi, i provvedimenti agricoli si devono compensare all'interno dei fondi dello stesso Ministero. Vice Ministro, non me ne voglia; ogni tanto convincete il Ministero dell'economia a dare qualcosa in più al settore agricolo, qualcosa che non sia da ritagliare in una sorta di guerra tra poveri all'interno delle varie componenti del settore agricolo.

(non volendo con questo gelare gli afflati, anche poetici, dei colleghi che mi hanno preceduto, in alcuni casi) non saranno i beneficiari - ove mai ve ne saranno - di questo provvedimento. Questo perché essi non sono professionali:

dovuto sottoporre ad un elenco tassativo dal punto di vista dei piani regolatori dei Comuni le zone dove dovrebbe essere proibito intervenire a estirpare gli alberi (gli agrumi, in questo caso).

coltivatori che, invece, continueranno ad essere colpiti dall'IMU agricola perché non sono professionali. Infatti, nella grande mistificazione dell'eliminazione dell'IMU in agricoltura abbiamo la piccola agricoltura tradizionale, limitando quella esenzione solamente agli agricoltori professionali. La maggior parte di coloro che con grande fatica tengono in vita gli agrumeti nei terrazzamenti, nelle zone costiere, nelle zone di collina, nelle zone delicate per il dissesto idrogeologico non sono professionali e, ancora una volta, non beneficeranno neanche di questo piccolissimo intervento. Io ero d'accordo con l'emendamento del senatore Puglia

assolutamente non operativo. Se poi tanto mi dà tanto, mi viene in mente l'ottima legge che approvammo la scorsa legislatura per la tutela degli alberi, che ancora non è stata applicata in tutto il Paese: questo provvedimento dovrà passare

quali e quanti di questi denari arriveranno veramente alla loro specifica destinazione, che poi - lo ripeto - già nel contenuto della legge non è una destinazione che privilegia l'agrumicoltura caratteristica tradizionale ma un ibrido tra questa e quella professionale. Per favore, non parliamo allora di politica agrumicola nazionale, perché in tal caso dovremmo parlare di interventi seri dovremmo parlare di blocco delle importazioni a seguito di trattati internazionali con Paesi che non fanno parte dell'Unione europea e che non sappiamo come producono (ma intanto arrivano comunque all'interno del nostro mercato) e dovremmo difendere le grandi produzioni; ma non è questo il contesto. Mi viene in mente, signor Presidente (forse lei era uno dei pochi presenti a quel tempo, o forse era alla Camera), quando, nel 1994, la senatrice Moltisanti si presentò in Aula con un'arancia, perché aveva trovato che alla *buvette* del Senato le spremute venivano fatte con arance con etichetta spagnola.

Avremmo potuto ricordare le lumìe pirandelliane, che forse non esistono più nel nostro panorama biologico caratteristico; saremmo dovuti scendere, secondo me, in particolari che invece questa legge - ahimè - non affronta.

del mandarino di Ciaculli a Palermo, che ormai esiste solamente nelle zone impervie di collina, perché per il resto, intervenire a favore della Conca d'oro significa difendere i condomini piuttosto che difendere gli antichi agrumeti che erano il vanto della Sicilia e di Palermo in particolare. Può darsi che questo disegno di legge solleciti e pungoli ad affrontare veramente il problema della agrumicoltura italiana, di quei 170.000 ettari di cui parlava il presidente Formigoni, che certamente non sono ricompresi nelle previsioni di questa legge. Quindi noi voteremo a favore.

tesoro dei contributi appassionati che sono venuti dalle senatrici del Partito Democratico, a testimonianza del fatto che il tema del paesaggio è un tema che non riguarda una Regione e che non riguarda un tipo di coltura. È un bene prezioso, che appartiene al Paese; infatti notavo che le senatrici intervenute sono una di Trieste, una della Toscana e una della Sicilia. Questo ha una valenza politica importante, che prescinde dalle dalle dimensioni del contributo e anche dall'accezione che in quest'Aula abbiamo sempre dato a questo tema quando abbiamo trattato la gran parte dei provvedimenti che riguardavano il settore agricolo.

pensiero lontana e di fatto arriva all'approvazione solo oggi, nonostante il travaglio che anche il Vice Ministro ha raccontato rispetto ad una legislatura che ha avuto nel proprio tragitto un cadenzario costante di provvedimenti dedicati al settore agricolo. Credo che siamo arrivati in fondo anche a questo provvedimento proprio perché questa è stata la legislatura che è riuscita a porre l'agricoltura nuovamente al centro e a riconoscere quello agricolo e agroalimentare come un settore non solo anticiclico, ma strategico per l'economia del nostro Paese. Con questo provvedimento, che pure si riferisce agli argomenti caratteristici e a una durata e a un intervento di tipo straordinario, si sancisce il legame definitivo tra l'agricoltura, il territorio e una storia che vogliamo riconoscere nel potenziale della tradizione, ma che si identifica anche

e proteggere quei luoghi significa non solo salvaguardare quanto di più bello offre il nostro Paese, ma anche avere rispetto nei confronti di chi continua ad abitarli ad abitarli ed avere responsabilità nei confronti delle future generazioni. Il paesaggio diventa quindi il risultato del passato, ma anche quello che vogliamo sia il nostro futuro. Ogni risultato parlamentare che si sia posto come obiettivo la tutela della biodiversità coincide con la capacità di saper coniugare oggi sviluppo e tradizione, sostenibilità dell'ambiente e crescita economica. La Convenzione europea sul paesaggio del 2000 fu sottoscritta a Firenze

un paesaggio da tutelare non solo con zone vincolate ma anche nel suo paesaggio agricolo, nelle zone urbane e nelle periferie. Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare agisce in un segmento del patrimonio paesaggistico, culturale e sociale

credo che dobbiamo essere molto obiettivi rispetto a una legislatura che aggiunge anche questi interventi ad una serie di altre misure che hanno lo stesso indirizzo. Ricordo, ad esempio, le risorse contro il dissesto idrogeologico e gli interventi in cui siamo intervenuti su settori molto specifici: gli uliveti, la viticoltura, il settore lattiero-caseario, il grano duro, l'ortofrutta, l'apicoltura e il miele, il settore florovivaistico.

del nostro Paese ad avere una sua centralità. Si tratta di scelte precise che stanno caratterizzando questo settore in modo innovativo innovativo e moderno, dove la sostenibilità deve stare insieme al rispetto della biodiversità e dove la tradizione diventa un elemento su cui costruire innovazione e sviluppo.

la necessità di sostenere e valorizzare un'agricoltura sempre più integrata, tradizionale e biologica sta diventando una vera priorità del comparto primario. il disegno di legge oggi in esame rappresenta l'espressione di questa tendenza per quanto riguarda gli agrumeti caratteristici. Sul punto, quando si parla di territorio d'origine, non si può prescindere dalle numerose aree agrumicole sparse in tutta Italia. Dal lago di Garda alla costiera amalfitana alla penisola sorrentina, passando per la Calabria e il Gargano, fino ad arrivare in Sicilia, l'intero Stivale vanta una diversità varietale che, però, non viene sufficientemente valorizzata. Con particolare attenzione al Gargano, c'è una diffusione a macchia di leopardo della coltivazione degli agrumi, con una superficie investita di circa 250 ettari. Vengono coltivate per lo più arance a polpa bionda, ma anche limoni e, in misura non troppo rilevante, mandarini. un territorio però che, purtroppo, ancora sconta l'ingente danno causato dall'alluvione del 2014, con tanti Comuni che tuttora navigano nell'incertezza e terreni afflitti da un sistema irriguo non al passo con i tempi. i tempi. Quando non sono le avversità atmosferiche a farla da padrone, pregiudicando gran parte dei raccolti, rimane la grande piaga delle tecniche di coltivazione arretrate, con potature saltuarie e concimazioni non soddisfattive alle reali necessità delle piante. A questo si aggiungono costi di produzione elevati, che penalizzano ulteriormente lo scenario ed espongono i pochi coltivatori rimasti a un distacco definitivo, stanchi di portare avanti un'attività che non cresce come dovrebbe. Arriviamo alle nostre proposte, credo di buon senso, che purtroppo non sono state accettate, come quella di ridurre i termini per l'emissione dei decreti attuativi del disegno di legge in parole. parole. Ad esempio, nell'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, nella definizione dei criteri e delle tipologie di interventi e nella determinazione dei contributi erogabili, abbiamo chiesto che i Ministeri interessati impieghino sessanta giorni e non novanta per emanare il decreto di riferimento. Al riguardo, ci siamo accorti, infatti, che dare troppo tempo all'Esecutivo equivale a disperderlo nel vuoto. Abbiamo anche chiesto che vi siano criteri ragionati nell'assegnazione dei contributi. Nello specifico, chiediamo che il contributo per gli interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici sia da attribuire prioritariamente non solo ai coltivatori e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, ma anche a particolari fasce deboli, come ha sottolineato prima anche il collega D'Alì: mi riferisco in particolare ai piccoli imprenditori agricoli e alle imprese a conduzione familiare e a chi ha terreni che ricadono nei territori dei Comuni che sono stati colpiti da eventi alluvionali, fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali. Lo stesso discorso va fatto anche per il contributo previsto a favore degli agrumeti caratteristici abbandonati, normato nell'articolo 4 Questo significa dare una boccata di ossigeno a quei territori che rischiano l'oblio e che altrimenti non riuscirebbero a riavviare seriamente l'attività colturale. Ancora, nelle procedure relative all'assegnazione dei contributi (articolo 7), il rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità deve rappresentare un passaggio obbligato. Abbiamo per questo chiesto che la graduatoria dei beneficiari, con l'indicazione dei fondi assegnati, sia pubblicata sul sito del MIPAAF, su quello della Regione di riferimento, oltre che dei Comuni interessati. Dov'è la trasparenza che tanto si auspica? Al fine di dare nuova linfa al settore, abbiamo chiesto che fossero previsti specifici benefici di carattere contributivo a favore delle imprese agricole che effettuano assunzioni di personale per l'espletamento degli interventi di ripristino degli agrumeti abbandonati.

che, seppure nelle sue imprecisioni e inesattezze, costituisce un primo passo verso la tutela di un ambito che rischia di essere soppiantato dalle produzioni massive e dalla allarmante concorrenza straniera; un quadro in cui, purtroppo, ci sono più ombre rispetto alle luci e dove la regola è data da una progressiva dismissione delle aree investite. Succede, infatti, che la combinazione di tecniche non innovative - da un lato - e interventi strutturali insufficienti - dall'altro - condanni la produzione di agrumi ai soli mercati locali. Per questo, concludo con un'esortazione chiara, che non lascia spazio a dubbi o interpretazioni. Basta *spot* e mancette: il comparto agricolo merita - secondo noi - molto di più.

Furono uccisi, in quella strage, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinari e Vito Schifani. Intorno all'albero Falcone, pochi minuti fa, hanno osservato un minuto di silenzio migliaia di giovani accorsi da tutta Italia che hanno fatto memoria, intorno a una dimensione progettuale educativa,

di Cosa Nostra con una condanna che riuscì a giungere fino a sentenza definitiva nel gennaio 1992, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nella sua Palermo, ha saputo rappresentare con parole chiare, ferme e decise,

proprio nei pressi di Capaci, nel luogo dove la voragine aperta fece tremare il Paese - sembrava un terremoto e fu una strage strage - è stata ricordata la Quarto Savona 15, la dizione con cui gli agenti di scorta si chiamavano. In quel luogo è stata finalmente collocata l'auto di scorta che, drammaticamente accartocciata, rappresentò allora il segno del dolore ma oggi è il segno della speranza, del cammino che, nel frattempo, il nostro Paese un Paese che via, via ha messo da parte il negazionismo della presenza delle mafie. Quante volte abbiamo potuto riscontrare questo atteggiamento devastante e corrosivo? Così come l'altro, forse più insidioso,

mafie, qualificandole però con tanti «però», che alla fine ci riporta proprio al negazionismo. Il Paese si è svegliato, ha fatto un cammino, ma ancora molto rimane da fare nella lotta alle mafie. Il Paese ha conosciuto una parziale verità della strage di Capaci; ha conosciuto le dinamiche interne a Cosa Nostra. Rimane ancora da scoprire il sistema delle collusioni,

quale caddero Paolo Borsellino, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina. Vorrei che non fossero mai dimenticate

Falcone, il 21 giugno 1989, caddero l'agente Nino Agostino, insieme alla moglie Ida Castelluccio, una donna che portava in grembo

è pronta a conoscere tutta la verità, anche la più amara e terribile, perché così un Paese diventa adulto e così possiamo guardare negli occhi le nuove generazioni, per camminare insieme a loro fino a liberarci dalla presenza delle mafie, di tutte le mafie.

forte dello Stato e a un'attività legislativa che ha rafforzato l'apparato di norme per contrastare ogni tipo di mafia, che proprio da quell'emergenza e da quelle ore drammatiche trasse una spinta decisiva.

nella facoltà di scienze politiche, facoltà di cui è stato anche preside dal 1980 al 1983. Con Papisca se ne va un punto di riferimento internazionale per i diritti umani e non solo. È una grande perdita: guida della facoltà di scienze politiche in anni non facili, fondatore del primo Centro universitario per i diritti umani in Europa, insignito del titolo di professore Jean Monnet *ad honorem* dalla Commissione europea. Con lui, il popolo della pace perde una delle sue guide più significative, uno dei suoi animatori più instancabili. I suoi insegnamenti e le sue lezioni sono stati il punto di riferimento del pacifismo politico cresciuto in Italia a partire dagli anni Ottanta, come non è accaduto in nessun'altra parte del mondo. Antonio era un uomo straordinario, tanto riservato da non ricorrere mai alla luce dei riflettori mediatici. Per questo motivo, molti non sanno quanto grande sia stato il suo contributo alla crescita nel nostro Paese di un'autentica cultura della pace. Antonio era uno studioso, un ricercatore e un intellettuale impegnato come pochi altri in quei movimenti della società italiana che generano cambiamento, partecipazione, impegno e trasformazione. Con Flavio Lotti, seduto accanto a padre Ernesto Balducci, il 15 marzo 1991 a Perugia ha lanciato la campagna per l'inserimento dell'articolo «Pace-diritti umani» negli Statuti degli enti locali e delle Regioni italiane. Antonio credeva fortemente nelle istituzioni e nella via istituzionale alla pace «Dal quartiere all'Onu» amava dire sempre - e descriveva efficacemente il campo d'azione dei costruttori di pace: dal piccolo al grande, dal locale al globale. Per questo, sin dagli anni Ottanta egli ha promosso l'impegno degli enti locali e delle Regioni per la pace e i diritti umani con una miriade di idee, campagne, documenti, proposte di legge, ordini del giorno, studi, rapporti e appelli,

Alla sua famiglia e a tutti coloro che con lui hanno lavorato e che ne sentiranno certamente la mancanza va un grande abbraccio dall'Assemblea del Senato.

venga in Aula a riferire sulle vicende che riguardano la scoperta di discariche abusive nell'area industriale di Cagliari. una questione che è sotto la valutazione della magistratura, la quale ha avviato delle indagini e scoperto gli illeciti. La magistratura ha proceduto e procede, con la nostra massima attenzione e fiducia, a verificare lo stato delle responsabilità proprio in ordine all'attività di un impianto industriale di trasformazione della fluorite - la Fluorsid - e alle modalità di stoccaggio e trattamento dei rifiuti industriali anche di natura tossica. Su questa indagine si è sviluppato un grande dibattito politico il Ministero è stato coinvolto in un'azione di indagine che riguarda l'area industriale di Cagliari, ma che probabilmente si potrebbe allargare alle altre aree industriali della Sardegna. Un tavolo permanente è stato costituito dalla Regione, dalle Città metropolitane e dai Comuni interessati. E grande è la preoccupazione, perché la gran parte delle aree industriali che ospitano siti di questa natura è limitrofa o addirittura ricomprende le zone umide della Sardegna, che sono delle vere e proprie oasi naturalistiche tutelate da convenzioni internazionali e di grande pregio anche ai fini dello sviluppo turistico e della valorizzazione ambientale delle risorse della Regione. Per questa ragione, signor Presidente,

Signor Presidente, intervengo su un argomento su cui ci sarebbe da piangere, ma forse è meglio che ci facciamo una risata.

Questo bravo uomo di novantacinque anni percepisce una pensione da reduce e una piccola quota da ex combattente. Ma ciò che non poterono né la guerra né la mina è riuscito a farlo la legge Fornero,

l'INPS e malgrado la Fornero».

circa una perdita del 50 per cento. Non abbiamo ancora le stime reali dei danni. È di oggi la notizia che le aziende di lavorazione hanno messo in cassa integrazione quasi tutti i dipendenti.

dunque preventivare, nelle prossime manovre finanziarie, una somma che oggi si stima, per difetto, in non meno di 30 milioni di euro, per dare una risposta e un ristoro a tutti gli agricoltori. Parlo della Provincia di Trento, ma la Provincia di Bolzano ha subito più o meno le stesse sorti. Può essere significativo - o non esserlo, visto che non ha una vocazione agricola - che l'Austria ha stimato 50 milioni di euro di danni agricoli derivanti dalle gelate. un invito al Governo a tenere in agenda questo episodio e a predisporre i giusti accantonamenti, perché bisognerà dare una risposta a un settore che ha subito una

per rispondere a un senatore. Presidente - come lei sa - un senatore, in base all'articolo 145, fa le interrogazioni al Ministro competente per avere informazioni e spiegazioni il Presidente, in base all'articolo 146, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dall'articolo precedente e non è formulata in termini sconvenienti,

stessi. Presidente, ho un fratello che è un pensionato e raccoglie i funghi e, quando li trova, li mangiamo assieme. Questo è il mio DNA familiare e ambientale. Forse altri hanno diversi DNA ambientali

e non i dipendenti, gli stipendiati, ovvero chi deve pensare a lavorare e a dare delle risposte